Comunico che in data 28 giugno 2013 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per la coesione territoriale:* «Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» comunico che in apertura della seduta pomeridiana di oggi sarà ricordata la figura di Margherita Hack. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,

LN-Aut e M5S).* Ma un Sottosegretario non ce l'hanno da mandarci? Non hanno un Sottosegretario disperso? Si sono dimenticati che questo è il Parlamento? Sono in giro a rinviare cose e non vengono in Parlamento? Parlamento? Presidente, sono veramente irritato, non sto facendo una sceneggiata. Lei sa, anche per le nostre storie precorse, che posso anche capire alcune situazioni,

lei incaricata di rappresentare il Governo. Tuttavia, pur non essendo lei direttamente responsabile, devo rappresentarle, perché sia riferito al Presidente del Consiglio e all'intero Governo, il gravissimo disagio del Senato, perché non può accadere, per rispetto del Senato e per la speditezza dei provvedimenti legislativi (tra l'altro si tratta della conversione di un decreto-legge che dovrebbe stare particolarmente a cuore al Governo), che il Senato sospenda i lavori per ben quaranta minuti a causa dell'assenza Quindi, la ringrazio per la disponibilità perché non ha nessuna colpa e, tuttavia, essendo lei parte del Governo, non posso esimermi dal sottolineare il disagio provato. Lo faremo anche formalmente, ma intanto credo di dover interpretare lo stato d'animo di tutti i colleghi che, forse, è ancora più forte

Sono testimone dell'impegno diretto della sottosegretario Vicari, di come ha seguito con costanza ed impegno l'esame del provvedimento in Commissione. Non altrettanto si può dire - purtroppo - di altri colleghi del Governo.

sui temi dell'efficienza e della prestazione energetica nel settore dell'edilizia. Richiamo velocemente (lascerò il testo integrale dell'intervento agli atti) i titoli di questa direttiva, i cui contenuti sono recepiti nel decreto-legge, a cominciare dall'adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, dalla fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli stessi e dall'introduzione, per la prima volta nel nostro Paese, di una definizione assolutamente fondamentale ed importante: quella dei cosiddetti edifici «ad energia quasi con conseguente redazione di una strategia nazionale per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale. Infine, ricordo l'adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici.

- hanno reso l'articolato indubbiamente più efficace e pregnante rispetto agli obiettivi richiamati. In questo senso va il ringraziamento a tutti i Gruppi per il lavoro e il contributo che hanno inteso dare. Il decreto contiene altresì, all'articolo 17, una norma che è una sorta di sanatoria rispetto alla classificazione degli installatori degli impianti da fonti rinnovabili. In una precedente norma infatti erano stati tagliati fuori alcuni di questi installatori, in particolare gli installatori artigiani; con il decreto-legge della cui conversione ci stiamo occupando viene sanata questa penalizzazione, ovviamente assolutamente inopportuna e da più parti lamentata, a cominciare dalle associazioni di settore, ma da tutti i Gruppi, anche con atti di sindacato ispettivo presentati negli scorsi mesi. Nella seconda parte del provvedimento - su questo mi permetto di soffermarmi brevemente - è inserita, in particolare all'articolo 14, la norma con cui si potenzia e si proroga l'attuale regime delle detrazioni fiscali del 55 per cento per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, prorogandone alla fine dell'anno la durata ed innalzando la quota di detrazione al 65 Vengono qui escluse dalle spese ammissibili a contributo quelle per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore.

All'articolo 16 è, invece, riportata la proroga al 31 dicembre 2013 del termine di scadenza (ora al 30 giugno 2013) dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF al 50 per cento prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare massimo complessivo ammissibile a contributo di 96.000 euro per unità immobiliare. La finalità della proroga è incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia con lo scopo di favorire sia la riqualificazione del patrimonio immobiliare del nostro Paese che la ripresa del mercato delle costruzioni, che rappresenta tradizionalmente uno dei comparti produttivi più importanti per la crescita del prodotto interno lordo nazionale.

che in Commissione ha avuto modo di fare il Governo, e cioè che l'importo di 10.000 euro va considerato aggiuntivo ai 96.000 relativi agli interventi edilizi. Si tratta di misure particolarmente importanti e in grado di contribuire a dare impulso all'edilizia specializzata in un Paese povero di materie prime come l'Italia. La nostra principale risorsa interna, infatti, è costituita proprio dall'efficienza energetica e dall'enorme conseguente possibilità di risparmio di positive ricadute in termini di abbattimento delle bollette dei consumatori. Per tali ragioni risulta fondamentale agire con determinazione e continuità sul patrimonio immobiliare, nonché sulla sua messa in sicurezza e sul suo efficientamento energetico. Tali misure in questi anni d'applicazione hanno rappresentato indubbiamente una delle principali azioni concrete di politica industriale adottate negli ultimi dieci anni, nonché uno degli interventi più significativi volti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali in campo energetico in vista del 2020. Il meccanismo delle detrazioni fiscali vincolato agli investimenti per la riqualificazione energetica e per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare ha fortemente convinto i consumatori: per l'estrema concretezza ed efficacia delle procedure e per l'automatismo che presiede all'erogazione dell'incentivo. Lo testimoniano i dati: nei primi cinque anni circa il 5,5 per cento del patrimonio edilizio nazionale è stato sottoposto a riqualificazione energetica; si stima che circa il 5 per cento delle famiglie italiane abbia usufruito di tali opportunità, per quasi 1,5 milioni di domande, con una previsione per l'anno in corso di altre 250.000 domande. Uno strumento utile, ancora, a sostenere la piccola e media impresa del nostro Paese, a valorizzare la filiera industriale italiana dell'edilizia e dell'impiantistica, contribuendo alla sua innovazione tecnologica, consentendo il mantenimento di livelli occupazionali e contribuendo alla emersione del sommerso in una fase cosi estremamente difficile per l'economia nazionale. A tutto ciò si aggiunga che tali misure hanno avuto ed hanno il pregio di smobilizzare una quota importante del risparmio interno verso iniziative produttive e dall'alto valore aggiunto.

per ovvi vincoli di bilancio, ovvero a individuare risorse, modalità e strumenti per stabilizzare, anche in forme diverse e più graduali, tali importanti incentivi dai risultati così decisivi. Al pari di questa e delle altre prima richiamate, restano ulteriori questioni controverse in questo testo rispetto alle quali sollecitiamo ulteriormente il Governo, come fatto nel corso dell'esame in Commissione, affinché anche nella discussione in Aula possano essere ricercate opportune sintesi: penso alla esplicitazione dell'ammissibilità agli incentivi richiamati degli interventi di messa in sicurezza degli edifici a rischio sismico e degli edifici di edilizia popolare (oggi esclusi) e alla delicata vicenda dell'aumento dell'IVA sui supporti integrativi ai prodotti editoriali, su cui condividiamo le preoccupazioni da più parte espresse. Si tratta, in conclusione, di un provvedimento importante e utile per il Paese in una fase così complicata e difficile. Auspichiamo possa essere ulteriormente migliorato anche nel corso di di questo passaggio parlamentare, che ovviamente riteniamo debba essere il più veloce possibile per dare ulteriore certezza agli investitori e alle famiglie. *relatore*. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli senatrici e senatori, il decreto-legge n. 63 contiene alcune disposizioni che propongono la proroga, ma con rilevanti modifiche, degli incentivi fiscali per il risparmio energetico nonché di quelli per le ristrutturazioni edilizie. Rammento che essi hanno origine lontane: dal 1988 per i *bonus* per le ristrutturazioni e dal 2007 per quelli per l'efficienza energetica. In particolare ecco alcuni dati a dimostrazione dell'importanza delle detrazioni fiscali per i comparti economici interessati: per le ristrutturazioni edilizie sono state presentate, a tutto il 2012, ben 5.470.000 domande, per un controvalore di opere di 94 miliardi di euro, con generazione di importi detraibili di 35 miliardi per i *bonus* per riqualificazione energetica, sempre al 31 dicembre 2012, le domande sono state 1.434.000 per opere d'importo pari a 17,2 miliardi di euro e importi detraibili per 9,4 miliardi di euro. Si tratta quindi di una manovra di tutto rispetto, la cui proroga oggi, nel pieno di una crisi che ha comportato una stasi significativa vari comparti, soprattutto in quello edilizio, potrà sicuramente dare respiro ai settori interessati. Va anche sottolineato che le procedure per ottenere le detrazioni a fronte di opere per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche hanno, come hanno avuto, un ulteriore effetto positivo: quello di consentire una maggiore trasparenza nei comparti interessati, con potere disincentivante per operazioni non fiscalmente regolari, tramite anche la necessità di validare i pagamenti tramite il cosiddetto bonifico parlante, e cioè quello contenente tutti i dati delle parti interessate (fruitore del *bonus,* impresa appaltatrice, codici fiscali e partita IVA,

con l'esclusione delle spese relative a pompe di calore ad alta efficienza e a impianti geotermici a bassa entropia e delle spese per la sostituzione di scalda acqua con apparecchi a pompa di calore. In pratica, vengono confermate come suscettibili di *bonus* le spese concernenti la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, il cambio d'infissi,

tetti massimi per le spese detraibili inferiori rispetto a quelli precedentemente in vigore, mentre restano confermati gli importi massimi delle detrazioni. La detrazione del 65 per cento è prorogata al 30 giugno

La detrazione è ripartita in dieci annualità di pari importo. Da segnalare infine che la detrazione convive con quella per le ristrutturazioni, ma le due agevolazioni non sono comulabili. La detrazione per il risparmio energetico compete altresì alle imprese, quand'anche costituite in forma societaria (società a responsabilità limitata, società per azioni ed altre), ma unicamente per interventi eseguiti

in misura pari al 50 per cento con un tetto massimo di 96.000 euro (a mio avviso per unità). Anche in questo caso la detrazione è ripartita in dieci annualità.

Le Commissioni riunite hanno, peraltro, accolto un emendamento che estende la predetta detrazione ai grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad

Gli articoli 19 e 20 dispongono, a partire dal 1° gennaio 2014, norme di natura fiscale per sopperire ai costi di cui alle precedenti disposizioni agevolative. L'articolo 19 prevede l'aumento dell'aliquota IVA al 21 per cento per i supporti integrativi allegati ai prodotti editoriali e precisamente: *gadget;* supporti integrativi (cioè CD o DVD) allegati alla rivista a scopo promozionale, ma senza alcuna diretta connessione con il prodotto editoriale; supporti funzionalmente connessi al prodotto editoriale quali, ad esempio, quelli allegati ai vocabolari, alle edizioni per la scuola le grammatiche delle lingue straniere che hanno scarsa operatività senza il connesso supporto che insegni la corretta pronuncia), i libri per l'infanzia, le pubblicazioni tecnico-professionali, eccetera. Al riguardo, ci auguriamo che il Governo accolga

L'articolo 20 dispone, sempre a partire dal 1° gennaio 2014, l'aumento dell'IVA dal 4 al 10 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate con distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cure, uffici, scuole, caserme ed altri uffici destinati a collettività. Con apposito emendamento le Commissioni riunite hanno proposto di estendere l'applicazione dell'IVA del 10 per cento alla somministrazione di alimenti e bevande effettuate tramite distributori automatici e, quindi, a tutte le somministrazioni, indipendentemente dal luogo di ubicazione dell'apparecchiatura. *(Applausi

Signora Presidente, signori del Governo, colleghi, il provvedimento che il Senato sta il Senato sta trattando contiene il recepimento della direttiva europea 2010/31/UE per mezzo di significative integrazioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ed altre importanti disposizioni (come abbiamo già sentito). Al di là della conferma, e contestuale incremento al 65 per cento, della detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica, sarebbe limitativo se ci trovassimo in presenza solo di un mero recepimento di direttiva atto ad evitare la prosecuzione della procedura di infrazione; potremmo, in tal caso, non riuscire a cogliere appieno un'importante occasione di rilancio. In questa prospettiva, vorrei brevemente riprendere il concetto di efficienza sviluppandolo in tre parti: l'efficienza energetica, l'efficienza economica e finanziaria, l'efficienza operativa. l'efficienza energetica, va sottolineata la necessità di promuovere azioni orientate al largo utilizzo di tecnologie *green* legate a materiali e sistemi di produzione italiana (si pensi soltanto alla mole di importazioni di legno, l'isolante termico per eccellenza per costruzioni, e alla connessa necessità di valorizzazione della filiera locale legno-energia) e insieme di promuovere azioni legate all'applicazione di dispositivi elettronici per il controllo in tempo reale di fabbisogno e consumo di energia dell'edificio, decisivi in termini di rapporto costi-benefìci, cogliendo inoltre l'occasione per promuovere il fondamentale raccordo tra risparmio energetico e divulgazione di tecnologie *smart,* da considerare con attenzione tra i presupposti per lo stesso ammodernamento digitale di cui alla specifica Agenda. In questa logica di integrazione tra tecnologie ed innovazione industriale, molto potrà fare il previsto piano di azione per edifici ad energia quasi zero (articolo 5), per il quale è auspicabile una riduzione dei tempi di predisposizione affinché pubbliche amministrazioni, progettisti ed operatori

Se ci si aspetta un articolato e sistematico riavvio di iniziative nel settore con prospettive ben più consistenti di quanto non possa riattivare solo la proroga delle detrazioni fiscali, allora la capacità di attivare forme di finanziamento non tradizionali rappresenta il possibile superamento di criticità. Ne cito soltanto due: il Patto di stabilità per gli enti pubblici e in generale l'accesso al finanziamento per pubblico e privato. In questa direzione auspico che trovi rapidissima definizione il contratto tipo che è stato demandato alla predisposizione dell'ENEA; che si intervenga per rendere il più semplice possibile l'intervento delle ESCO; che si attivi una verifica di efficacia ed utilizzo del mercato dei titoli di efficienza energetica. Efficienza economica significa infine ottimale utilizzo del danaro: va sottolineata anche in questo caso l'esigenza che le indicazioni del disegno di legge, molto puntuali, si traducano in criteri di priorità per l'attribuzione di sostegni ed incentivi pubblici nel nome della spesa efficace, capace cioè di attivare efficienza con 1'occhio al rapporto investimento su energia risparmiata. Infine, vi è l'efficienza operativa. Questo ambito riguarda la filiera di azioni da far procedere in modo coordinato ed operativo ed include la ricerca, la formazione, la produzione, conclusione, è necessario attivare in concreto, tra 1'altro, le diverse articolazioni dell'efficienza affinché divengano anello anello di congiunzione tra 1'esigenza di ammodernamento tecnologico del patrimonio immobiliare privato e pubblico, divengano supporto e stimolo alla ricerca al progresso tecnologico dell'industria,

gli obiettivi del disegno di legge in ordine al risparmio energetico divengano «sistema». Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge oggi all'esame di quest'Aula (il cosiddetto "decreto ecobonus") si prefigge la finalità di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità a quanto previsto dalla legislazione comunitaria. L'introduzione di misure di sostegno a politiche volte a promuovere l'efficienza energetica e, in generale, di misure per lo sviluppo sostenibile rappresenta senza dubbio un'importante spinta ed un passo avanti verso la ripresa dell'economia e del rilancio dei consumi. Tra i punti più qualificanti del decreto la previsione di edifici a energia quasi zero; ancora, le norme in tema di proroga degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e la relativa estensione all'acquisto di arredi. In particolare, le misure relative alle detrazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, oltre che prorogare le disposizioni già in vigore, prevedono un forte potenziamento, come ricordato, dell'attuale regime di detrazioni, che passerà dal 55 per cento, per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, al 65

con una significativa riduzione dei costi, contribuendo in tal modo al rilancio dei consumi e ridando contestualmente vitalità a tutto il settore edilizio e delle aziende dell'indotto, che da tempo vive grandi difficoltà. Proprio in edilizia si registra una rivoluzione progettuale, tecnica e costruttiva, fondata sulla rapidità, la sicurezza e la sostenibilità ambientale, cui non si assisteva da decenni. Un settore fondamentale (rappresenta il 10 per cento del PIL in Italia), sul quale intervenire promuovendo un'opera di rigenerazione urbana che consenta il risanamento su vasta scala di intere aree delle città e dei territori. L'azione di riqualificazione abitativa del patrimonio esistente punta a migliorarne il *comfort* e ad introdurre nelle costruzioni concetti di sostenibilità energetica ed ambientale; il tutto nel rispetto del territorio, che va custodito e non violentato. Mi permetto di sottolineare l'importanza che nel decreto assume la detrazione per le spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Il decreto riconosce, infatti, tale detrazione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un massimo di 10.000 euro. hanno lavorato intensamente per cercare di migliorare il provvedimento e correggere il tiro su alcuni degli aspetti più dibattuti. Per quanto riguarda il tema delle detrazioni è stata prevista l'estensione del beneficio per i mobili anche agli elettrodomestici (prima non contemplati), anche a libera installazione, di classe non inferiore alla «+». Non da ultimo leggiamo, in questi giorni, con grande preoccupazione, dei fatti succeduti alla presentazione del piano industriale della nota azienda Indesit. L'insieme di queste disposizioni potrebbe contribuire in maniera significativa a restituire vitalità ad un settore cruciale della manifattura italiana come quello del legno arredo, che da alcuni anni vive una profonda crisi, soprattutto nel Centro Italia, con conseguenti e gravissime ricadute occupazionali. Nel corso dell'esame in Commissione abbiamo tentato, con diverse proposte, di estendere ulteriormente i benefici previsti. Tuttavia, abbiamo dovuto contemperare le esigenze di rilancio del settore con i vincoli di bilancio e la ristrettezza delle risorse e adottare le soluzioni più equilibrate, considerati tutti i fattori e le esigenze in gioco, sia in termini di crescita che di tenuta del sistema. In particolare, si è cercato di introdurre un'ulteriore proroga dei tempi e di alzare il tetto di spesa previsto, soprattutto a seguito dell'estensione del beneficio agli elettrodomestici. Appare infatti problematica l'inclusione degli elettrodomestici, seppur giusta, senza ampliamento del tetto previsto, in quanto tale inclusione va a comprimere gli effetti stessi attesi dal provvedimento sulla spesa per i mobili. È necessario sul punto un impegno concreto del Governo affinché si reperiscano le risorse necessarie ad una reale ripresa dell'economia, consentendo soprattutto alle piccole e piccolissime imprese di rimettersi in gioco. In tal senso l'impegno prossimo del Governo dovrebbe essere orientato a prorogare la scadenza prevista al 31 dicembre 2013, ad aumentare i tetti di spesa previsti e ad individuare le misure necessarie ad estendere il meccanismo della detrazione anche ad altri settori della manifattura italiana. Occupazione e sviluppo economico sono una priorità per tutto il Parlamento. Ogni misura, a nostro avviso, deve premiare il saper fare, l'impresa diffusa e il lavoro, per ridare dignità per ridare dignità al nostro Paese. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, nella prima parte del decreto, gli articoli da 1 a 13 recepiscono la direttiva UE n. 31 del 2010, apportando modifiche puntuali al decreto legislativo n. 192 del 2005. Con questo, seppur tardivo, recepimento della direttiva eviteremo che la Corte di giustizia europea applichi le sanzioni economiche connesse alla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della suddetta direttiva. Certo, evidenziamo come impropria la scelta del Governo di intervenire in materia attraverso lo strumento del decreto-legge, visto che gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza energetica sono di natura ordinamentale. Nell'articolato in questione, infatti, non si riscontrano carattere di necessità ed urgenza e dunque sarebbe stato giusto intervenire con un decreto legislativo. Ma comprendiamo, di ulteriori sanzioni non ne abbiamo bisogno, ci bastano e avanzano quelle pesanti e umilianti inflitte nei giorni scorsi dalla Corte di giustizia europea per i ritardi cronici nella realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti della Regione Campania. La seconda parte del decreto cerca di rispondere alle attese dei contribuenti e delle imprese che operano nel mercato immobiliare. Si occupa delle detrazioni, delle disposizioni finanziarie e della qualificazione degli installatori. Il regime di detrazione fiscale viene prorogato per sei mesi, sino al 31 dicembre 2013, sia per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, innalzando l'ecobonus dal 55 al 65 per cento, sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Novità importante, non solo per gli immobili privati oggetto di ristrutturazione, viene introdotta per la prima volta l'agevolazione fiscale per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all'arredo, seppur calcolata su un ammontare complessivo di spesa limitato a soli 10.000 euro. Anche questa è un'azione importante che darà sostegno alle imprese che operano nel settore. Peccato però che la somma non si aggiunge al massimale di spesa di 96.000 euro ma è inclusa. Analizzando in dettaglio alcune disposizioni tecniche del provvedimento, come Gruppo Lega Nord riteniamo importante l'introduzione, all'articolo 5, del concetto di «edifici ad energia quasi zero», in riferimento agli edifici di nuova costruzione delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 31 dicembre 2018. Obbligo che però non può che passare da un'esclusione delle spese d'investimento dei Comuni dal Patto di stabilità. Abbiamo invece più di una riserva per le previsioni dell'articolo 6 che disciplina il rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici pubblici e di quelli privati non solo in caso di costruzione, ristrutturazione e compravendita, ma anche in previsione di nuova locazione dell'edificio. Appare chiaro che l'introduzione dell'obbligo di rilascio di tale attestato comporterà inevitabilmente, da un lato, un aumento dei prezzi degli immobili e, dall'altro, maggiori costi a carico degli affittuari, che si affiancheranno ai pesanti rincari dei canoni derivanti dall'oneroso passaggio nel 2012 dall'ICI all'IMU del Governo Monti, votata da PD, PdL e UDC. Altre pesanti incombenze, introdotte sempre dall'articolo 6, riguardano ad esempio i ridottissimi tempi per le pubbliche amministrazioni per dotare gli edifici dell'attestato di prestazione energetica. Tempi che rischiano di non essere rispettati. Per Comuni e Province significa, a PEG 2013 approvato, trovare non poche risorse e affidare gli incarichi velocemente. Anche la validità decennale dell'attestato, pure in assenza di intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell'edificio, ci sembra eccessiva. Il Gruppo della Lega Nord vede invece favorevolmente gli articoli del decreto che introducono proroghe al regime di agevolazione fiscale. Tali agevolazioni rappresentano un valido strumento di supporto agli investimenti delle imprese dell'edilizia e dell'indotto, a sostegno della loro crescita e del loro sviluppo. I positivi effetti di tali misure ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo contribuiscono all'emersione del sommerso

chiediamo che venga applicato il massimo rigore contro i furbi chiedendo l'annullamento dei benefici fiscali in caso di accertamento di immobile abusivo, non in regola con il pagamento dell'IMU. Infine, un'osservazione che ritengo debba far riflettere i colleghi e soprattutto coloro che in tema di risparmio energetico sono mossi da ansie di prestazione. La prima parte del decreto-legge recepisce la direttiva europea che, se da un lato rappresenta un impulso e favorisce la sensibilità in tema di interventi di risparmio energetico, dall'altro comporta ulteriori incombenze e oneri per la pubblica amministrazione e i contribuenti. È per questo che sarebbe opportuno evitare di fare i primi della classe andando oltre le richieste della direttiva europea, visto il periodo di crisi economica. In questo senso, l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e accolto dalla maggioranza in Commissione, che pone l'obbligo dell'attestato anche in caso di trasferimento di immobile a titolo gratuito, non lo condividiamo assolutamente e vi voteremo contro. Cittadini del Senato, buongiorno. Noi siamo un Paese per definizione industrializzato ed energivoro. La nostra bolletta energetica nazionale incide sulla bilancia commerciale per cifre spaventose, destinate ad aumentare. Nonostante questo, noi ci comportiamo come se fossimo ricchi produttori arabi o texani del tempo che fu. Infatti ci permettiamo di sprecare energia con disinvoltura, come se questo non avesse alcun peso sulle sorti del nostro Paese. Qualche settimana fa ha destato scalpore la notizia che una domenica pomeriggio questo Paese si sia alimentato a costo zero per un paio d'ore, grazie alle energie rinnovabili. Si è gridato al miracolo e si è detto che questa è la strada: produrre energia pulita, riducendo il costo della bolletta energetica nazionale e riducendo anche la nostra dipendenza dalle fonti fossili, di cui notoriamente non abbiamo grande disponibilità. Tutto vero, per carità, ma questa è solo una parte della soluzione. Occorre infatti lavorare per aumentare l'efficienza energetica. In Europa, come al solito, ci sono arrivati prima di noi. In Germania, ad esempio, hanno capito che occorre utilizzare l'energia nel modo migliore, nell'industria, nei trasporti, nell'agricoltura, nelle infrastrutture e nelle case. E mentre in Germania, come in Svezia e in molti altri Paesi, si implementa la capacità di garantire un determinato processo produttivo o l'erogazione di un servizio (ad esempio il riscaldamento) attraverso l'utilizzo della minor quantità di energia possibile, in Italia si preferisce rispolverare il nucleare o l'energia prodotta dall'incenerimento dei rifiuti indifferenziati, da affiancare alle fonti rinnovabili, forse per tacitare le coscienze. Ma davvero pensiamo di poter riempire d'acqua uno scolapasta? Pensiamo che le energie rinnovabili siano l'unica soluzione? Occorre cambiare prospettiva. Vogliamo ricordare a noi tutti che l'energia è il grande *dominus* dello sviluppo e della trasformazione per come l'abbiamo concepito nell'era capitalistica; un'era destinata a finire. In un momento in cui la disponibilità delle fonti fossili a basso costo è in crisi irreversibile, è indispensabile percorrere la strada che ci porterà alla decarbonatazione della produzione e del ciclo di vita. Rendere efficiente un sistema significa fare in modo che possa funzionare con una minore quantità di energia e che sia energia proveniente da fonti di qualità, cioè prodotta anch'essa in modo efficiente e senza incidere sull'ambiente. Dobbiamo intervenire, quindi, non soltanto sull'offerta di energia, ma anche sulla domanda. Non pensate che si tratti di ridurre semplicemente i consumi, di risparmiare. Risparmio ed efficienza non sono sinonimi: con l'efficienza si risparmia, ma non è sempre vero il contrario. Dobbiamo fare di più utilizzando meno energia. Pensate soltanto alle ricadute in termini occupazionali che un'efficace campagna di efficientamento produce. Pensate anche soltanto alla riqualificazione del nostro (immenso) patrimonio edilizio. Le nostre imprese edili, che soffrono la crisi forse più che altrove, devono (sottolineo devono) trovare nella riqualificazione la strada per risollevarsi. (sottolineo devono) rinascere a nuova vita e diventare un modello da imitare. Potremmo persino combattere la tendenza, tragica, al consumo del territorio, evitando di costruire nuove abitazioni, di cui non abbiamo bisogno, ma riqualificando l'esistente, adeguandolo ai parametri dell'efficienza energetica. Cari colleghi, oggi abbiamo una grande opportunità e una grande responsabilità: dobbiamo programmare, pianificare e realizzare strumenti operativi e strategie che permettano di consumare meno energia a parità di servizi offerti e dobbiamo farlo con lungimiranza, guardando ai prossimi cinquant'anni e non alla prossima settimana. In quanto a capacità di programmare, purtroppo, questo Governo e quest'Aula non si sono dimostrati all'altezza delle aspettative fino ad oggi. È infatti ancora vivo il ricordo delle infinite proroghe e dei tanti, troppi commissari nominati negli ultimi mesi per l'ansia di «fare» a qualunque costo qualsiasi cosa, senza costrutto. Per questo, colleghi, diamo una prova di maturità, non solo oggi, ma anche in seguito, evitando che gli interessi delle *lobby* e la burocrazia vi «costringano» in futuro a rinviare, modificare o abbandonare questa che è la strada più logica, quella che sceglierebbe un buon padre di famiglia. Vedrete che chi verrà dopo di noi ce ne sarà grato. Grazie signori del Governo, onorevoli colleghi, il tema dell'efficienza energetica e della riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano può e deve rivestire, nell'ambito delle politiche economiche che il Governo intende perseguire, un ruolo prioritario, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nelle costruzioni sono misure importanti al fine di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e per ridurre le emissioni di gas responsabili dell'effetto serra. È anche il momento in cui conviene osservare, con attenzione ancora maggiore del solito, l'economia del nostro Paese, perché il nostro sistema produttivo è stato colpito da una crisi mondiale senza precedenti che ha acuito le difficoltà storiche del sistema imprenditoriale italiano, un sistema articolato e complesso, oggi non fertile all'iniziativa industriale e, ancor di più, alla *green economy*. La linea portata avanti dal Governo con il provvedimento in esame evidenzia lo sforzo dell'Esecutivo nell'impegno, obbligatorio, verso l'Europa per due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, ma offre anche la possibilità di intervenire per favorire lo sviluppo e promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico di settori vitali per l'economia quali quello energetico e quello ambientale. Il potenziamento dell'attuale regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, anche alla luce degli emendamenti presentati, darà sicuramente un forte impulso all'economia di settore e in particolare al comparto dell'edilizia specializzata, un settore caratterizzato da una forte base occupazionale, concorrendo in questo momento di crisi al rilancio della crescita e dell'occupazione e allo sviluppo di un comparto strategico per la crescita sostenibile. Ritengo opportuno, onorevoli colleghi, consentire la possibilità di ricorrere in maniera più efficace a questi strumenti incentivanti in favore di famiglie e imprese, prevedendo l'opportunità di ricorrere ad opere di demolizione e ricostruzione con piccoli aumenti di volumetria; una possibilità improntata chiaramente al rispetto delle normative ambientali, collegata al raggiungimento delle più alte classi energetiche al fine di anticipare gli *standard* europei e attivare una serie di numerosi piccoli interventi che possono offrire occasioni lavorative per la piccola imprenditoria locale. Tutto questo può essere una base su cui costruire una politica energetica che consenta a tutti gli edifici di nuova costruzione, entro il 31 dicembre 2020, di essere a energia quasi zero. È necessario, dunque, intervenire con questo provvedimento non solo per rispondere direttamente a disposizioni europee, ma anche per cogliere l'opportunità di innescare nuovi processi di sviluppo che garantiscano crescita economica e sostenibile. e sostenibile. A fronte dei maggiori adempimenti amministrativi che la stessa direttiva europea prevede per le amministrazioni pubbliche, chiamate a svolgere un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica, è altresì apprezzabile l'introduzione di misure volte a ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle pubbliche amministrazioni. Anche le Regioni dovrebbero adeguarsi a questo nuovo sistema costruzioni prevedendo, nella prossima programmazione regionale integrata a quella comunitaria 2014-2020, interventi collegati anche e soprattutto alla luce dell'avanzamento di strumenti operativi di trasformazione delle città. Si guardi, ad esempio, al piano città, in grado di favorire le politiche urbane attraverso l'affermazione della rigenerazione urbana e ambientale come chiave strategica per lo sviluppo. Occorre implementare politiche di sviluppo urbano intelligente che evitino il collasso di un territorio, come quello italiano, già fortemente compromesso. compromesso. Ma è necessario favorire, altresì, il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in quanto risorsa da tutelare anche ai fini di prevenzione dei rischi idrogeologici.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, ringrazio il senatore Tomaselli per il lavoro Grazie sul tema dell'*energy retrofitting*, ossia della riqualificazione energetica, che cercano di cogliere la sostanza delle questioni riportate nel decreto-legge Per una serie di ragioni l'attenzione nei confronti del patrimonio immobiliare si è notevolmente sviluppata. Si è trattato di un processo lungo, che ha seguito, com'è naturale, un percorso culturale che ha generato una consapevolezza diffusa su temi che hanno il loro centro nella qualità del costruire, nella sicurezza sismica, nei consumi energetici, nel risparmio idrico, nei materiali edilizi, nel *comfort* degli ambienti. purtroppo non è avvenuto che alla fine di un potente ciclo economico che ha poggiato saldamente sullo sviluppo edilizio. L'industria delle costruzioni ha sempre sostenuto le fasi di sviluppo, ma negli ultimi vent'anni è stata anche protagonista di bolle speculative e finanziarie che hanno addirittura reso tumultuosa l'espansione urbanistica ed edilizia. Oggi ci troviamo quindi con un cospicuo patrimonio edilizio le cui caratteristiche sono spesso insufficienti, specialmente riguardo alle prestazioni energetiche. Per essere chiari, non sono solo gli edifici realizzati nel secondo dopoguerra ad avere basse prestazioni energetiche: anche l'edificato progettato nei primi anni 2000 alcune volte non ha caratteristiche molto migliori.

si capisce l'importanza della riqualificazione, che oggi è prima di tutto una riqualificazione energetica e un miglioramento antisismico. del patrimonio edilizio esistente è stata ormai sviscerata in molte delle sue implicazioni tecniche, ed è possibile fare alcune sintetiche considerazioni, che potranno sembrare elementari,

la parte preponderante delle superfici disperdenti, l'intervento sull'involucro determina il più forte recupero di prestazioni. Il secondo intervento è sull'impiantistica, in particolare sui generatori di calore e sui sistemi di termoregolazione degli ambienti. Su questi due punti principali va va a convergere sostanzialmente l'intervento di riqualificazione che dà la sostanza del risparmio edilizio nella riqualificazione del patrimonio costruito. fare la riqualificazione energetica? In molti si pongono questa domanda, ed innanzitutto occorre definire rispetto a cosa va misurata la convenienza. Qui si entra in un terreno delicato, perché determinate scelte possono essere ritenute giuste e quindi necessarie a tutti i costi; diversamente, analizzare i costi, invece, consente di avere alcune indicazioni utili. Da verifiche che ormai sullo storico sono state approfondite, anche con studi di università o nell'ambito di progetti europei che mettono a confronto le esperienze in vari Paesi dell'Unione, emerge che gli investimenti mediamente investimenti mediamente plausibili, che sono quelli che ricordavo prima, cioè gli interventi sull'involucro e sull'impiantistica, hanno tempi di ritorno (*payback period*) che si aggirano intorno ai venti anni. *payback period* di questo tipo sono scarsamente appetibili, anche per una famiglia che possa ritenere di aver comprato l'abitazione della vita. Investimenti che hanno questa lunghezza di ritorno si calcolano pensando pensando di pareggiare l'investimento con i risparmi attesi sulle bollette energetiche degli anni che verranno. A questo punto, si coglie il perché degli incentivi: se non diamo gli incentivi, non facciamo tornare i tempi di ritorno in termini accettabili, che scendono appunto a dieci anni, consentendo anche forme di finanziamento che possono essere attivate. dà la possibilità ai cittadini che comprano o anche che prendono in affitto un immobile di fare una scelta non solamente rispetto ai criteri che a loro più interessano, ma anche rispetto ad un tema preciso. Quindi, portare avanti l'attestato di prestazione energetica sia per

sovraccarichi di regolazione rispetto a quella minima dalle fonti comunitarie», in particolare ad «evitare di introdurre o di mantenere adempimenti (...) non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive». La fonte di questa definizione è sul sito del Governo italiano. Ora, ci troviamo in sede di conversione di un decreto che si prefigge l'obiettivo di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili, sostenere la diversificazione energetica, promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico e conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

Nell'articolo 21 invece, al comma 1, si provvede ad incrementare, nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ai commi 2 e 3, si provvede al rifinanziamento del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi nel 2008. In particolare, viene rifinanziato l'articolo 5 della legge n. 7 del 2009 per ben 413 milioni di euro per il periodo 2014-2023, al fine di reintegrare le risorse necessarie all'attuazione della legge di ratifica citata, ovvero per la realizzazione di iniziative speciali a beneficio del popolo libico, nonché la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina ed altresì per la realizzazione di progetti infrastrutturali di base che vengono concordati tra i due Paesi. non so chi tra i miei colleghi qui presenti conosce particolari di attuazione in merito a questo Trattato Italia-Libia, però forse l'ho trovato io (lo dico con estrema ironia) il nesso della collocazione in questo decreto del rifinanziamento di questo Trattato Italia-Libia: il nesso sia l'articolo 18 del Trattato, denominato «Collaborazione energetica», cioè una norma sostanzialmente pro ENI, visto che la norma praticamente prevede il rafforzamento del partenariato in tale settore attribuisce particolare rilievo alle energie rinnovabili, incoraggiando la cooperazione tra enti ed organismi dei due Paesi, sia sul piano industriale su quello della ricerca e della formazione. Ma il punto specifico è il seguente: nell'articolo 21 si devono rilevare diversi aspetti problematici in relazione alle modalità utilizzate per la copertura finanziaria del decreto-legge in esame, soprattutto con riferimento alle disposizioni che rifinanziano gli interventi della legge di ratifica del Trattato con la Libia e, successivamente, riducono a copertura gli stessi stanziamenti recati dal medesimo Trattato. Si tratta di un'operazione contabile molto poco chiara. Si rappresenta, infatti, che, trattandosi di risorse in conto capitale, il loro utilizzo per finalità di natura corrente (minori entrate correnti) rappresenta una dequalificazione della spesa. Andrebbe poi chiarito più puntualmente l'impatto sull'indebitamento pubblico. Inoltre, si fa presente che le risorse in questione sono finalizzate all'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con il Trattato di amicizia con la Libia stipulato nel 2008: adempimento che lo storno delle relative risorse sembrerebbe rendere inevitabile rinviare. Appare infine evidente una cospicua insufficienza della copertura per circa 368 milioni di euro, in rapporto al 2024, in violazione al comma 3 dell'articolo 17 della vigente legge di contabilità, che impone la puntuale indicazione della copertura, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme. Dalla norme. Dalla relazione tecnica si evince che le risorse utilizzate a copertura per 229 milioni di euro sarebbero insufficienti anche soltanto alla copertura dell'autorizzazione di spesa di 413 milioni di euro. I cittadini del Movimento, alla luce del fatto che parte cospicua degli oneri è configurata come previsione di spesa, evidenziano la necessità di corredare la clausola di copertura di apposita clausola di salvaguardia. Pertanto, crediamo sia il caso di inserirla.

il decreto-legge n. 63 si pone, tra i principali obiettivi, quelli di migliorare la prestazione energetica degli edifici, promuovere la competitività tecnologica dell'industria e conseguire gli obiettivi nazionali in materia di energia. Il provvedimento sostiene concretamente le famiglie che affrontano la ristrutturazione di un immobile. Grazie alla proroga e all'aumento delle detrazioni è più facile perseguire gli obiettivi di efficienza energetica previsti dalla direttiva del 2010 del Parlamento e del Consiglio europeo. È proprio con questo spirito che, sottoscrivendo una lettera, lo scorso 10 maggio 34 senatori di tre forze politiche di maggioranza, tutte le associazioni imprenditoriali, industriali, artigianali e commerciali del settore e le tre principali organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno chiesto al Ministro dello sviluppo economico l'ampliamento delle agevolazioni anche a settori complementari alle ristrutturazioni ed in particolare a quello del legno arredo e a quello degli elettrodomestici. fatto che il decreto ricomprende esplicitamente i mobili, congiuntamente ad altri senatori abbiamo presentato un emendamento per estendere la detraibilità anche ai grandi elettrodomestici bianchi di libera installazione e in classe energetica efficiente. Detto emendamento ha trovato il parere favorevole delle Commissioni bilancio, finanza e industria e del Governo ivi rappresentato. L'unanime convenire si spiega con il convincimento che i cittadini possano godere di maggiori agevolazioni senza che queste gravino sui conti pubblici, visto che non è stato modificato il limite di 10.000 euro già previsto nel decreto per i soli arredamenti. Oltre ad aiutare le famiglie, si dà un'opportunità all'industria degli elettrodomestici, che vanta una bilancia commerciale attiva in quanto da sempre siamo un Paese esportatore. La nostra industria, peraltro, continua a sostenere con propri finanziamenti l'innovazione tecnologica, con una rilevante attività di ricerca e sviluppo, al fine di creare prodotti con prestazioni energetiche sempre più efficienti. Non solo la manifattura, ma anche il commercio del settore rappresenta un fiore all'occhiello del Paese: poche multinazionali e moltissimi imprenditori italiani, le cui imprese offrono un servizio qualificato al consumatore, anche grazie al continuo ammodernamento dei punti di vendita e alla formazione del personale. Nella sola distribuzione al dettaglio trovano occupazione 24.000 lavoratori,

Il comparto sviluppo ha un giro di affari di circa 10 miliardi di euro, di cui oltre un quinto generato dagli elettrodomestici, settore che, dal 2011 ad oggi, in solo due anni e qualche mese, ha perso il 19 per cento del fatturato. In conclusione, signor Presidente, estendere gli ecobonus ai grandi elettrodomestici bianchi di libera installazione e ad alta efficienza energetica significa mantenere viva la ricerca per l'efficientamento dei consumi energetici, garantire un elevato livello di occupazione, specialmente di quella giovanile, sostenere i consumi interni oggi pesantemente depressi, aiutare concretamente le famiglie italiane che vogliono investire nella casa per il loro futuro. *(Applausi dal

A questo provvedimento abbiamo presentato alcuni emendamenti e due ordini del giorno per provare a migliorarlo ulteriormente, per provare a mettere in luce due questioni che, credo, vadano affrontate.

che consente di usufruire dei benefici per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico alle sole società che investono queste detrazioni e usano questi benefici per edifici dedicati esclusivamente alla produzione. Questa è un'interpretazione molto restrittiva, che impedisce a una parte importante dell'edilizia sociale di questo Paese di intervenire per ristrutturare i propri alloggi. Penso alle cooperative a proprietà indivisa, alle 40.000 famiglie che abitano nei relativi alloggi, dove i residenti non hanno titolo per ristrutturare, e quindi non hanno la possibilità di beneficiare di queste detrazioni, detrazioni, ma, dall'altra parte, alla proprietà cooperativa non viene riconosciuta la possibilità di godere di questi benefici.

possibilità di consumare meno, appare veramente un'utopia rispetto alla condizione di tanti quartieri popolari nelle nostre grandi città. Giustamente questo provvedimento sottolinea la necessità di dare una priorità alle sedi della pubblica amministrazione, alle scuole, per interventi di efficientamento energetico. Noi pensiamo che anche il patrimonio pubblico vada nominato, che ci sia bisogno di un intervento serio su un patrimonio pubblico tanto degradato, su cui è necessario intervenire innanzitutto nell'interesse degli abitanti, della qualità della loro vita, nonché dei nonché dei costi che gli abitanti delle case popolari devono sostenere di fronte a spese che in assenza di un'efficientamento energetico sono sempre più alte. Ma è anche interesse pubblico fermare il degrado, per non svalutare ulteriormente un patrimonio grande come quello dell'edilizia residenziale pubblica. Mi auguro che il Governo e questo Parlamento, in sede di esame degli emendamenti, dedichino attenzione a questi temi.

le potenzialità del nostro Paese su un versante delicato, come la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in una prospettiva di conformità alla normativa europea e nella piena consapevolezza degli obblighi da questi previsti. Non va dimenticato, tra l'altro, che siffatte disposizioni hanno una priorità inderogabile: quella di coniugare in maniera pragmatica tre aspetti, sostenibilità, crescita ed occupazione, linee operative che dovrebbero essere il riferimento indiscusso dell'azione di Governo e di qualsivoglia intervento, soprattutto in una fase tanto delicata per il Paese in cui alcuni comparti operativi sono praticamente fermi. I rappresentanti delle maggiori categorie di settore hanno evidenziato anche, nelle audizioni svolte in Commissione, la loro soddisfazione nei confronti del provvedimento. Com'è stato da loro sottolineato, il decreto-legge può avere effetti positivi sull'economia italiana, intervenendo a sostegno di un settore particolarmente rilevante che al momento vive una forte *impasse* operativa. Si faceva anche riferimento ad alcuni studi che confermerebbero il grande potenziale, con un ritorno economico positivo, di molti interventi di efficienza energetica previsti dal provvedimento, sebbene - a mio avviso - non adeguatamente approfonditi. Dinanzi a queste esigenze inderogabili, il Parlamento avrebbe dovuto avere come priorità quella di elaborare modalità di intervento efficienti e pragmatiche, capaci di travalicare i limiti della politica, il peso degli interessi e puntare diritto all'efficienza di una norma e alla sua rapida esecuzione. Ma purtroppo così non è stato. Non possiamo trascurare l'assenza di una risposta univoca del Governo dinanzi al generale rafforzamento e potenziamento delle formule incentivanti adottate. Così come non possiamo trascurare le dinamiche alquanto discutibili che hanno contraddistinto lo svolgimento dell'*iter* legislativo del provvedimento stesso, a partire dalle Commissioni di competenza alle quali è stata assegnata il decreto in sede referente. Le complessive finalità del decreto-legge e l'esame dei singoli articoli hanno attestato una competenza piena e primaria della Commissione ambiente, che avrebbe potuto esprimersi secondo modalità più rispondenti alle sue competenze specifiche.

si allontana dalle potenzialità inespresse che la mancata sede referente ha determinato. A ciò si aggiunge il fatto che poi le osservazioni e le condizioni da questa espresse non sono state minimamente tenute in considerazione dalle Commissioni in sede referente. Appare discutibile a questo punto accettare che una Commissione, seppur competente nello specifico per oltre il 70 per cento del provvedimento, debba limitare la propria operatività e ridimensionare il proprio margine di intervento, magari accettando supinamente quanto indicato dal Governo o quanto emerge negli accordi discutibili che ci sono stati. Tutto questo ci spinge a riflessioni più complesse, soprattutto alla luce di quanto è andato poi delineandosi presso le Commissioni in sede referente, dove i rappresentanti del Governo hanno mostrato non poca rigidità e chiusura e dove le scelte emendative al decreto-legge sembrano essere state dettate non dal confronto o dall'approfondimento su determinate questioni, ma da opportunità di natura politica. Appare lecito chiedersi di cosa dovrebbe, dunque, occuparsi una Commissione. Nel caso della Commissione bilancio probabilmente la priorità è stata quella di formulare pareri di natura politica che andassero a sostituire quelli di natura finanziaria a cui essa dovrebbe essere tenuta. Sicuramente non hanno lasciato indifferenti i pareri negativi dati dalla Commissione bilancio ad alcune proposte di emendamento che, malgrado non recassero alcun onere, sono state estromesse dal confronto e dalla discussione per ragioni che ci sfuggono. L'elevato numero di pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rende necessario un approfondimento di natura politica per quegli aspetti che non sono strettamente afferenti alla valutazione sull'adeguatezza della copertura finanziaria. Un esempio alquanto chiaro può essere offerto da un emendamento, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere negativo, all'articolo 2 del decreto-legge che introduce una rinnovata definizione di cogenerazione con il rischio di creare criticità e poco funzionali duplicazioni di quanto già esistente. Sebbene l'emendamento prevedesse l'utilizzo di definizioni già previste da direttive comunitarie e da norme nazionali di recepimento, prevedendo la definizione di cogenerazione e di cogenerazione ad alto rendimento attraverso l'esplicito richiamo dei riferimenti normativi, è stato bollato come oneroso. A tal riguardo sarebbe opportuno che la Commissione bilancio ci spiegasse i parametri entro i quali è chiamata ad operare e quali sono i criteri in base ai quali provvede ad escludere una proposta di rettifica dal confronto parlamentare. Non intendo esprimere criticità circa le dinamiche politiche che spesso sottendono le scelte e che protendono verso l'accoglimento di questa o quella proposta di emendamento. Ma ritengo che i due versanti (quello tecnico-finanziario e quello politico) debbano mantenersi ben separati o, almeno, avvicendarsi nelle sedi che a queste sono deputate. La promiscuità di questi due versanti o la loro reciprocità rischiano di inficiare in maniera vistosa la *ratio* stessa dell'agire parlamentare e del confronto democratico alla base dell'*iter* legislativo. L'atteggiamento conflittuale tra alcuni referenti di Governo e parlamentari a cui abbiamo assistito in Commissione si traduce nell'incapacità di avere un approccio strategico univoco verso il decreto-legge, mortificando di fatto il ruolo del Parlamento e riducendolo alla sola presenza. Il decreto-legge Il decreto-legge dovrebbe servire a rilanciare alcuni comparti economici garantendo, nel contempo, l'efficienza energetica, ma in questo modo si limita all'osso il margine di intervento, rimandando ancora una volta le misure reali per cause di natura politica. Quanto accaduto rappresenta una metafora della funzionalità operativa di questo Parlamento in merito alla quale invito tutti i presenti a riflettere. Abbiamo offerto la possibilità di apportare correttivi in una prospettiva di crescita e di efficienza, ma non c'è stata data l'opportunità di contribuire a migliorare il provvedimento. Faccio riferimento alle proposte di emendamento finalizzate ad evitare nuove procedure di infrazione, sollecitando il testuale recepimento degli articoli 6 e 7 della direttiva 2010/31/UE. Sarebbe stato strategico per l'attuazione del piano casa, degli interventi di ristrutturazione urbanistica e del piano per le città inserire letteralmente la previsione normativa della direttiva in ordine all'adozione di sistemi alternativi, tra cui la cogenerazione. Un ulteriore richiamo va fatto alle definizioni novellate dall'articolo 2, comma 1, tra le quali sarebbe stato opportuno, al fine di evitare confusioni ed errate interpretazioni, inserire la definizione di fonti rinnovabili integrata da quella di biomassa più aggiornata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Sarebbe stato il caso di operare in maniera armonica e coerente con quanto previsto già dalla normativa, al fine di non creare quelle conflittualità tali da legittimare un'*impasse* operativa. Ma c'è chi «ci marcia» nella confusione normativa. Sarebbe stato ulteriormente opportuno intervenire sull'articolo 14, ampliando la platea degli interventi destinatari di formule incentivanti, ad esempio, attraverso la previsione dell'utilizzo incentivato delle pompe di calore nell'ambito della produzione efficiente di energia e, ad esempio, attraverso unità ed impianti di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento negli edifici che garantiscono la produzione efficiente di energia. Questa, a mio avviso, si sarebbe potuta inquadrare come una volontà di intervento ad ampio spettro che, garantendo il recepimento di quanto disposto dalla direttiva n. 2010/31/UE, ha ha l'obiettivo primario di rimettere in moto l'economia dando lavoro ad aziende e incrementando i livelli di efficienza. che dobbiamo rimettere al centro il ruolo del Parlamento. La congiuntura economica, le difficoltà del Paese e l'urgenza di essere celeri non possono e non devono essere usate come scusanti per bypassare i normali *step* di confronto parlamentare. Questo è un dovere nei confronti dei cittadini che attendono da noi le risposte. Il mio obiettivo è quello di spostare il confronto degli emendamenti dalla Commissione all'Aula. Pertanto, non ritirerò quelli a anzi avrò cura di intervenire su ognuno di loro proprio per farne comprendere la portata ed avviare un ragionamento costruttivo in una sede che a questo sarebbe deputata, se non altro fino a quando non percepirò un po' di buon senso.

63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. La decretazione d'urgenza si rende necessaria per evitare al nostro Paese pesanti sanzioni per non avere rispettato gli obblighi della direttiva n. 31 del 2010 dell'Unione europea, che - ricordo - è volta a promuovere la prestazione energetica degli edifici, delle loro parti e delle unità immobiliari per favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea e all'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici. Gli obiettivi del decreto-legge in esame sono volti a promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, a sostenere la diversificazione energetica e a rendere competitiva l'industria italiana con lo sviluppo tecnologico. I vantaggi che si otterranno con questo decreto, anche alla luce di alcune modifiche al testo apportate nelle Commissioni riunite 6a e 10a, riguardano le detrazioni fiscali sugli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Si passa - appunto - dal 55 per cento al 65 per cento. L'aumento di percentuale della detrazione potrà sicuramente ridare impulso all'economia del settore e soprattutto al comparto dell'edilizia specializzata, che fornisce alti livelli occupazionali. Nel merito, spetterà la detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese documentate e sostenute a partire dal 1° luglio 2013 sino al 31 dicembre 2013 e al 30 giugno 2014 per le ristrutturazioni importanti dell'intero edificio. Ancora, entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere ad energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018. Viene previsto un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici, che comprende informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato è obbligatoria in caso di costruzione, vendita o locazione di un edificio o di una unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla pubblica Il fondo di garanzia è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento della efficienza energetica nell'edilizia pubblica. Inoltre, gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a importanti ristrutturazioni sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Si prevede, inoltre, l'estensione dello sconto IRPEF del 50 per cento per mobili finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, ai grandi elettrodomestici, anche a libera installazione, di classe non inferiore alla A per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. L'estensione del *bonus* ristrutturazione è riferita ai soli elettrodomestici da incasso. I proprietari di immobili che stanno effettuando, o che effettueranno, ristrutturazioni immobiliari potranno dunque usufruire di uno sconto IRPEF del 50 per un ammontare non superiore ai 96.000 euro fino alla fine dell'anno e, dentro questo limite, una quota di 10.000 euro può destinata all'acquisto di mobili a partire dal 1° luglio. Con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività, l'emendamento a mia firma apporta correzioni alla norma al fine di rendere chiaro che le suddette somministrazioni, in qualsiasi luogo e forma effettuate, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 mi auguro che il decreto-legge in esame possa essere convertito al più presto dall'Aula, proprio in virtù di quanto accennato nelle premesse, e cioè che è necessario ed urgente favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del nostro patrimonio immobiliare in conformità alla direttiva europea del 2010.

Presidente, quello che successe la sera del 29 giugno 2009 a Viareggio è qualcosa di inimmaginabile: 33 persone persero la vita in maniera assurda, mentre in una tranquilla serata estiva stavano stavano passeggiando, guardando la televisione o tornando a casa. Le domande di risarcimento presentate per il sostegno finanziario dopo l'incidente sono state 127, ma solo 101 sono state accolte. Da portavoce dei cittadini, ho raccolto il messaggio dello scrittore Gianluca Ferrara, che mi appresto a leggervi: «Oggi, 29 giugno, sono trascorsi quattro anni dalla strage di Viareggio. Una strage in cui sono state uccise 33 persone da una criminale mentalità che tutela il capitale lasciando il lavoro privo di sicurezza. Il mandante, è bene ricordarlo, è questo modello economico. Mauro Moretti, l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, definì la strage "uno spiacevolissimo episodio". Una frase che infanga la memoria di chi è stato vittima e acuisce il dolore dei superstiti e dei familiari delle vittime. Una giustizia perseguita dal macchinista Riccardo Antonini che gratuitamente ha messo a disposizione dei familiari delle vittime la sua consulenza e per questo è stato licenziato. Sono trascorsi quattro anni da quel maledetto 29 giugno e in via Ponchielli (la strada distrutta dal fuoco) i lavori devono ancora terminare. Lo spazio antistante la strada fino a tre giorni fa era completamente invaso da erbacce che rendevano la zona degradata e abbandonata, ma pochi giorni prima di ogni 29 giugno come ogni anno, in poche ore, ripulito il tutto. Intanto sulla casina dei ricordi dove sono conservati i messaggi, le immagini di quella terribile notte d'estate, la bandiera del nostro Paese sventola ancora a mezz'asta. Verrà alzata solo quando ci sarà giustizia». In attesa di verità e giustizia, chiedo alla Presidenza che, nella prossima seduta, per lo meno quest'Aula mantenga vivo il ricordo dedicando alle vittime un minuto di silenzio. Signora Presidente, come ricordava la senatrice Bottici, sono trascorsi ormai quattro anni da quella tragica notte e quattro anni sono tanti, ma non per Viareggio, non per chi ha perso gli affetti più cari, non per una città che fa fatica ad uscire da un incubo che si è portato via 32 vite, seminando distruzione e sgomento, terrore e dolore. Le case sono state ricostruite, ma le ferite dell'anima e del cuore non si possono ricucire. Per questo, signora Presidente, la ringrazio a nome di tutti i familiari e dell'intera città se consentirà di ricordare con un minuto di silenzio in quest'Aula quella notte d'inferno, perché proprio in questo momento abbiamo più bisogno che mai della vostra solidarietà, della vostra vicinanza. Siamo infatti nel bel mezzo di un'udienza preliminare presso il tribunale di Lucca che, come ricorda Daniela Rombi, presidente dell'associazione che riunisce i familiari delle 32 vittime, è molto lunga e dolorosa. Durante questa udienza a tutti noi, e purtroppo ai familiari, è toccato ascoltare assurdità vergognose che aggiungono dolore su dolore, sgomento e rabbia. Un avvocato difensore dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, ha detto nell'aula del tribunale di Lucca che il disastro era prevedibile perché l'infrastruttura è piena di elementi che possono aprire un carro, disfare una boccola, sfondare una cisterna. E proprio in questo momento, in cui si sta svolgendo l'udienza preliminare, un altro avvocato di Ferrovie ha appena spiegato che 32 morti bruciati non sono una strage ma una disgrazia; disgrazie che, ascoltando ancora gli avvocati di Ferrovie, si possono ripetere ogni giorno perché - così si argomenta - la rete ferroviaria non è un biliardo e ci sono un'infinità di elementi che possono aprire un carro, sfondare una cisterna. Questo ascoltano i familiari delle vittime, i feriti, chi piange lutti e distruzioni. Ma Viareggio è tornata in piazza e si è stretta attorno ai suoi morti e alla richiesta di verità e giustizia che non può non trovare risposta. Infatti, se oggi è tempo di lutto è anche tempo di speranza. Ho fiducia nella giustizia e nella possibilità concreta di ottenere le risposte implorate in questi anni. Tradire questa fiducia, che è quella di un'intera città e, mi auguro, di un intero Paese, sarebbe come assegnare un colpo mortale a chi crede che almeno la giustizia possa dare un po' di pace a chi avrà per sempre la vita sconvolta da una tragedia troppo grande. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).* Signora Presidente, a nome del Gruppo del Popolo della Libertà mi associo alla richiesta di un momento di ricordo particolare della strage di Viareggio. Mi associo anche nel considerare con non grande favore quanto accaduto dopo, soprattutto in ordine alle lungaggini

Vorrei che in futuro queste cose non accadessero più, e soprattutto che non accadesse che ogni volta, per ottenere una risposta celere da parte delle autorità competenti, siano esse amministrative che giudiziarie, si debbano creare associazioni di familiari e si debba spingere attraverso i mezzi di comunicazione. E questo per ottenere risultati che in un Paese civile dovrebbero arrivare tempestivamente. Credo che il vero risultato positivo di questa azione dovrebbe essere quello di avere la certezza, che nel campo della prevenzione di questi incidenti, il nostro Paese abbia fatto dei passi avanti; che, sull'onda

legittimo e assolutamente condivisibile di ottenere giustizia vera, sarebbe anche quello di avere un risultato forte in ordine alla struttura della modernità del nostro Paese, in maniera tale che questi episodi non abbiano mai più a verificarsi.

e aggiungiamo pochissime considerazioni. Intanto aspettiamo tutti, insieme con i cittadini di Viareggio, il momento della verità. L'inchiesta ha già dimostrato che, al di là delle responsabilità personali, esiste un problema serio di manutenzione e di messa in sicurezza generale della rete ferroviaria per il trasporto delle merci e per la rete dei pendolari. il migliore contributo che da queste Aule parlamentari possa venire alla lotta per la verità dei cittadini di Viareggio sia trovare anche le risorse necessarie per porre fine a questa continua precarietà delle nostre reti ferroviarie. Non possiamo pensare di trovare soldi solo per investire in opere faraoniche per l'alta velocità

chiediamo - è ci aggiungiamo alle richieste accorate fatte - verità e giustizia per la strage di Viareggio, che non è soltanto la strage della città di Viareggio, ma una delle più orrende stragi che ha colpito noi cittadini italiani.

al cordoglio profondo e commosso per la commemorazione di quel terribile giorno in cui si è consumata a Viareggio, in tutto il Paese, una tragedia inaccettabile. Oltre a ringraziare anche per la concessione che verrà fatta di commemorare con un minuto di silenzio in quest'Aula questa terribile tragedia, vorrei aggiungere l'auspicio che questo silenzio si interrompa per una chiarezza e una verità che è stata anche da altri invocata. Chi conosce personalmente quella zona, quella viabilità ferroviaria, forse ha il sospetto fondato, insieme a tutte le famiglie coinvolte, che quella tragedia potesse essere evitata. Quattro anni sono tanti per non essere riusciti ad arrivare a un approfondimento: vogliamo augurarci che si cominci a lavorare per arrivare ad una verità che riporti giustizia e assicuri una condizione di prevenzione di altri disastri, ormai inaccettabili in un Paese moderno e avanzato. Signora Presidente, ovviamente anche noi del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà condividiamo quanto è stato detto su questa strage prevedibile, ma crediamo che un minuto di silenzio non basti. Dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto (e ringrazio la collega Bottici di averci ricordato Bottici di averci ricordato questa tragedia), dalla senatrice Petraglia e al senatore D'Alì, sono arrivate grandi accuse al capo indiscusso, il padrone, di Ferrovie dello Stato da qualche decennio, ossia Mauro Moretti. Credo che giustizia sarà fatta quando quest'Aula concretamente chiederà con una mozione che si dimetta perché inadeguato a guidare Ferrovie dello Stato. Colleghi, nell'associarmi al cordoglio e al ricordo delle vittime della strage di Viareggio, rappresenterò al Presidente la richiesta, che sicuramente sarà accolta, di

ma abbiamo letto con allarme le dichiarazioni della professoressa Lorenza Carlassare sui lavori per la modifica dei Titoli della Carta costituzionale. Oggi siamo ancora più allarmati e ci chiediamo cosa stia succedendo, cosa, al di là delle parole, accadrà alla nostra Costituzione ora che apprendiamo dai mezzi d'informazione che J.P. Morgan, colosso finanziario *leader* nei servizi globali, in un rapporto sulla crisi dell'euro del 28 maggio scorso afferma che in Europa non si riescono ad applicare le necessarie misure di *austerity* a causa delle Costituzioni antifasciste, Costituzioni con Governi deboli rispetto ai Parlamenti si legge - deboli nei confronti delle Regioni, dei lavoratori e dei loro diritti; Costituzioni che prevedono la licenza di protestare se sono proposte modifiche sgradite. che quella che si era creduta una crisi solo economica è invece una crisi anche politica, dovuta al fatto che le Costituzioni dei Paesi del Sud dell'Europa (Spagna, Italia e Grecia) sono nate a seguito della caduta di regimi fascisti sull'onda dell'entusiasmo liberale e democratico e per questo pongono un limite politico alle manovre di *austerity* e all'integrazione europea, che altro non è che cessione di sovranità nazionale. La relazione continua invitando per questo motivo, con il chiaro intento di continuare più massicciamente con le misure di *austerity,* i Paesi mediterranei a liberarsi delle proprie Costituzioni antifasciste. Ricordiamo a noi stessi che l'opinione di J.P. Morgan non è l'opinione di un privato cittadino qualunque, perché tale istituto conta quasi un migliaio di banche di credito ordinario, banche d'affari e *holding* in tutto il mondo. Alla luce di tutto ciò ci chiediamo e chiediamo al Governo in che considerazione tiene queste affermazioni e se esse influiranno e in che modo sulla riforma della nostra Carta costituzionale.

non era poi così difficile. Sarebbe bastato ricordarsi la dura reazione alle dichiarazioni rilasciate solo sei mesi prima nel corso di una conferenza stampa ad Aversa, in provincia di Caserta, dal suo predecessore, Renato Balduzzi, perché il neoministro della salute Beatrice Lorenzin, cogliendo un'ottima occasione per restare in silenzio, evitasse non solo l'indignazione dei comitati e delle associazioni che da anni lottano per la difesa dell'ambiente in cui vivono (o meglio, sopravvivono), ma soprattutto l'ennesima grave offesa ad una popolazione che da anni ormai vede i nomi dei propri cari affollare le liste ospedaliere dei malati di tumore e sempre più spesso anche i necrologi di questi territori. Il ministro Lorenzin riconosce che vi è un'impennata dei tumori nelle persone che abitano nei territori che insistono lungo il confine tra le province di Napoli e Caserta, peccato che affermi che la causa dipenda dagli stili di vita della gente. Forse però il Ministro non sa che la gente che abita in questo territorio, che per motivi che non vogliamo ricordare è stato ribattezzato «terra dei veleni», oggi sta provando a migliorarlo quello stile di vita, e lo fa mangiando proprio i prodotti genuini, i prodotti della propria terra. È una terra che da secoli regala a questo territorio e a tutto il Paese eccellenze assolute in campo agroalimentare, come le rinomate fragole di Parete, la mozzarella dei Mazzoni, la mela annurca giuglianese, per non dire altro; lo sta migliorando aumentando l'attività fisica, attraverso l'utilizzo sempre maggiore delle biciclette, dato comprovato dall'aumento delle vendite in questo settore. Qualcosa allora non quadra. Se la gente mangia sano e fa tanto sport, come mai in questo stesso territorio anno dopo anno le statistiche continuano a parlare di incrementi vertiginosi di patologie tumorali, malformazioni fetali, gravi infezioni delle vie respiratorie, e tanto altro ancora, che inondano le liste dei presidi ospedalieri e sempre più spesso anche le liste dei necrologi? Forse la gente non sa che molti di quegli eccezionali prodotti che consuma con tanto orgoglio provengono da alcune terre piene zeppe delle sostanze altamente tossiche che negli anni della famosa emergenza rifiuti hanno hanno viaggiato in maniera occulta lungo l'asse Nord-Sud, finendo dritte dritte nelle nostre campagne e di conseguenza sulle tavole di tutta Italia. Ma forse la gente sa fin troppo bene tutto ciò, per questo poi si indigna così tanto quando un Ministro della Repubblica, che sicuramente queste cose non le sa, viene a prenderli in giro fino in casa propria con la solita storiella della mancanza del nesso di causalità tra inquinamento da rifiuti ed effetti sulla salute, il cui unico scopo, molto probabilmente, è quello di voler coprire - ribadisco, coprire - ad ogni costo una verità che, se ufficialmente riconosciuta, darebbe il via a una spirale risarcitoria inimmaginabile. Signora Presidente, cari colleghi, celebriamo in queste ore l'ingresso della Croazia nell'Unione europea e il presidente Napolitano ha rappresentato tutti gli italiani a Zagabria. È un momento storico per quel Paese, ma è soprattutto un'ottima notizia per l'Europa tutta. ciò ci regali un rinnovato entusiasmo nel progetto comunitario e ci dice, in un tempo di eurofatica quando non di aperto euroscetticismo, che non si è spento il mito fondativo dell'Unione, il fascino che ancora esercita sui popoli europei, il sogno dei nostri padri (di Schumann, De Gasperi, Adenauer, Spinelli), quello di un processo che ha dato il via all'area più sviluppata del mondo, i cui membri hanno conosciuto il più lungo periodo di pace e di benessere della storia. testimonia - lasciatemelo dire - che la strategia dell'allargamento da parte dell'Unione Europea è stata di straordinario successo, capace di forzare positivamente il cambiamento di aree strategiche nel nostro continente: l'ingresso della Croazia ricuce infatti ferite che scavano in profondità nella storia europea. Si tratta di un evento che avrà forse effetti modesti a Bruxelles, ma è un fatto politico fondamentale in vista del definitivo aggancio dei Paesi dei Balcani, che appartenevano all'ex Iugoslavia, all'orbita europea. Lasciatemi dire che questa portata storica è percepita ancora più come un fatto importante per chi, come me, viene da una terra, quella del confine italiano nordorientale, che ha sofferto tristemente le tragedie del Novecento. Non voglio dimenticare coloro che hanno dovuto abbandonare le proprie terre, ma lasciatemi ricordare oggi - lo faccio credo a nome di tutto il Senato - le comunità italiane che

ricordando il ruolo dell'Italia, che dobbiamo esprimere attraverso due direttrici. La prima è nei confronti della Croazia: siamo il primo *partner* commerciale e dobbiamo rimanerlo; dobbiamo rafforzare i progetti di collaborazione e cooperazione attraverso l'Iniziativa centroeuropea e l'Iniziativa Ma è importante che il nostro Paese sia in prima linea per portare a termine il processo di integrazione di tutti i Balcani occidentali. I sei anni di negoziati che hanno portato all'ingresso della Croazia nell'Unione europea sono stati eccessivamente lunghi. Ora le nuove sfide si chiamano Serbia e Montenegro,

Signora Presidente, colleghi, stamattina in provincia di Varese, nel Comune di Cardano al Campo, è avvenuto un fatto gravissimo:

accettabile che possano succedere fatti di questo genere ad amministratori che sono il punto di riferimento dei loro cittadini, sono il presidio della legalità e dell'ordine nel loro territorio. La persona che ha sparato è un ex dipendente, o comunque un dipendente sospeso,

venendo meno quella solidarietà che deve legare una comunità intera. Per quanto si possa pensare ad un atto barbaro di una persona che può aver perso il bene dell'intelletto in un certo momento, dobbiamo comunque tenere alta la tensione e l'attenzione per quanto sta accadendo. Vorrei anche ricordare che Laura Prati è una donna che sul territorio si è sempre battuta per i più deboli e soprattutto per i diritti delle donne; in un'iniziativa proprio riguardo al femminicidio ed è sintomatico che sia stata colpita la prima donna diventata sindaco a Cardano al Campo. In tale contesto vorrei davvero che le senatrici

La Presidenza e l'intero Senato si associano agli auguri ed alla solidarietà per questi amministratori, nonché alle preoccupazioni da lei espresse su quello che sta avvenendo nel Paese. **Sul 20° anniversario Signora Presidente, voglio richiamare l'attenzione di quest'Aula su una data importante di cui oggi si ricorda il ventesimo anniversario. Era il 2 luglio 1993 e nella battaglia del Checkpoint Pasta a Mogadiscio morirono tre nostri militari e 36 furono i feriti

vogliamo ricordare chi, al servizio dello Stato, ha sacrificato la sua vita per il rispetto della libertà e la tutela della pace fuori e dentro i confini nazionali.